ratifica un'intesa sindacale che realizza importanti risultati sul terreno della previdenza e del precariato:

qualche passo in avanti nei contratti a termine contenuti nella legge Maroni sul mercato del lavoro. Si tratta, dunque, di un momento importante e di un provvedimento importante su un'intesa sindacale che ha avuto un rilievo non marginale. Eppure, ho la sensazione che siamo arrivati a questo appuntamento attraverso un percorso che non soddisfa sia nel metodo sia nei contenuti.

con la quale guidare l'intesa tra le parti. È vero che esisteva a monte il programma il programma con il quale il Governo si è presentato alle elezioni e le ha vinte ed è vero che questo programma conteneva gli elementi fondamentali della trattativa (parlava del superamento dello scalone della legge Maroni, del superamento della legge Maroni sul mercato del lavoro, della necessità di intervenire

non era chiaro - o almeno a me non è apparso chiaro - che ci fosse una volontà esplicita da parte dell'Esecutivo di realizzare, con le parti sociali, quei punti fondamentali del il popolo italiano aveva espresso il suo consenso al momento delle elezioni. Questo ha portato ad una situazione nella quale non sono apparsi con grande precisione gli obiettivi che il Governo si proponeva e tutto è stato rimesso al contraddittorio tra le parti sociali. Devo dire che anche su questo terreno, mentre è stata martellante l'iniziativa della Confindustria, peraltro significativamente accompagnata da un coro di opinione pubblica ad essa favorevole, non altrettanto importante mi è parsa l'iniziativa da parte del sindacato. Non è compito mio decidere su questo e dare un giudizio. Certo è che in una trattativa che aveva i caratteri di cui ho parlato e che in qualche maniera richiedeva un'azione sindacale decisa, a me non è parso che questa sia stata supportata dalla necessaria mobilitazione. È stata una scelta non la voglio discutere, ma mi resta l'impressione che se si fosse spinto di più da parte delle organizzazioni sindacali, si sarebbe potuto ottenere di più. C'è stata poi la consultazione dei lavoratori, una consultazione molto ampia. Non la definirei un *referendum*, intanto per l'ostilità al *referendum* sugli accordi e sui contratti sindacali espressa negli anni, e anche recentemente, da almeno una delle confederazioni. Se si sta dalla parte del *referendum* sugli accordi - e io sono da questa parte - ci si sta sempre: ci si sta sempre: negli accordi aziendali, nei contratti di lavoro e nelle grandi consultazioni; non si può scegliere il terreno sul quale fare democrazia sindacale.

per diluire nel tempo il superamento dello scalone dovevano essere riequilibrati all'interno dello stesso sistema previdenziale, ha fatto sì che questi costi, tolti per i lavoratori che si trovavano immediatamente di fronte allo scalone, vengano redistribuiti nel tempo a svantaggio dei lavoratori che andranno successivamente in quiescenza.

osservatori: è vero che è stata introdotta la cosiddetta quota per la realizzazione del momento in cui si può andare in pensione, con una combinazione di anzianità di servizio e di anzianità di lavoro, ma

Non c'è dubbio che se la caratteristica del lavoro usurante è l'acquisizione di un diritto soggettivo, perché i lavoratori sottoposti all'usura sono tutti i uguali, non si capisce come mai per alcuni di essi saranno garantite, con le risorse messe a disposizione,

questione è quella dell'esigibilità effettiva di un rapporto tra salario e pensione non inferiore al 60 per cento per coloro che oggi sono giovani e che matureranno la loro indennità previdenziale tra molti anni. caso l'accordo non è chiaro; anzi, direi che è proprio uno dei punti più oscuri dove andavano e vanno fatte delle precisazioni per trasformare delle clausole puramente enunciative di un diritto in effettività esigibilità. Così come ci sono misure non sufficienti sul superamento della continua ripetizione iterativa dei rapporti di lavoro a termine.

non riescono o possono non riuscire a superare la forza della norma. In ogni caso, si vede che non c'è un limite forte alla prosecuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

connesso con questo stato di disoccupazione. Ebbene, piuttosto che questo, dice Maroni nella sua legge, si preferisce avere un miglioramento di questa condizione introducendo come lavoro parzialmente trasparente quello che prima era lavoro nero. E però questo non viene realizzato in sovrappiù, alla condizione normale, ma a detrimento delle condizioni costituite come condizioni forti. È quindi vero che c'è un miglioramento della qualità della disoccupazione, ma vi è anche un peggioramento della qualità dell'occupazione. Ora, poiché queste cose sono emerse con forza anche nel dibattito sindacale, io credo che il contributo del dibattito in Parlamento doveva, poteva portare ad un inquadramento giuridico più forte di quello contenuto nell'intesa (che intesa era e non contratto di lavoro) e tutti sanno che le intese si realizzano anche sulla base di compromessi, dove l'ambiguità e l'equivoco recitano un ruolo fondamentale tra le parti. Quindi, trasformando questo in una norma, era necessario dare a questa un contenuto, un inquadramento giuridico più forte. A quel punto è emersa una concezione della concertazione tra le parti sociali e col Governo come un sistema di intese chiuse e immodificabili. ora la seguente osservazione. Se gli accordi con le parti sociali sono stipulati come canoni su cui ricalcare strettamente le leggi, essi assumono un valore di fonte normativa. Le stesse organizzazioni sociali assumono una configurazione di soggetto legislatore e dunque di soggetto politico in senso stretto. Si tratta di una concezione che io non esito a giudicare di carattere neocorporativo, implicazioni sull'assetto istituzionale e sul sistema politico. Ne segue un problema: quale sarebbe la legittimazione esplicita dei soggetti sociali a compiere questo ruolo? Quali princìpi costituzionali applichiamo ai soggetti sociali per fare eseguire loro con certezza questo ruolo? Come si risolve il problema del monopolio della rappresentanza politica del mondo del lavoro che in tal caso verrebbe sussunta dai movimenti sindacali? Come si risolve il problema dello spiazzamento delle forze che appartengono al grande filone italiano ed europeo del lavorismo? Se non rispondiamo a questi problemi - e non lo facciamo, nella circostanza di questa intesa e della sua traduzione in norma - la crisi dell'autonomia oggettiva del sindacato dalla politica si fa strada, e si fa strada anche una crisi altrettanto pericolosa: quella dell'autonomia delle forze politiche e delle forze sociali. Aggiungo che alcune voci sindacali non le nomino ma le riconoscerete - sono state spiacevolmente cacofoniche con il nostro impianto costituzionale. Il Parlamento non scrive leggi sotto dettatura. Il punto è così decisivo per oggi e per domani che meriterebbe da solo il rifiuto del Protocollo a prescindere dal merito dell'intesa. Ho sentito argomenti diversi esposti qui dal senatore Larizza ma non sono convincenti. C'è il problema della garanzia dell'intesa tra Governo e parti sociali: questa garanzia il Governo la formula quando stende il testo conclusivo del Protocollo trasformato in norma, non può impedire o evitare che avvengano modifiche o addirittura miglioramenti del testo. Se poi si vuole l'intangibilità, allora il Governo ponga sul piatto della bilancia se stesso: ponga la fiducia, che è l'unico strumento per fare questo. Se ci sarà la fiducia sul Protocollo, anch'io la voterò; se non ci sarà la fiducia, mi esprimerò nel voto come quelli consultati dal sindacato e che nella misura del 25-30 per cento hanno detto che non erano d'accordo e volevano modifiche al Protocollo. Anch'io voglio queste modifiche: se ci sarà la fiducia la voterò, se non ci sarà la fiducia seguiterò a battermi perché queste modifiche si realizzino.

una coincidenza questa discussione così rilevante sulla condizione di lavoro e sulla fine di una vita di lavoro per milioni di lavoratrici e lavoratori nel Paese giorno dei funerali degli operai morti a Torino, in cui il Senato è doverosamente presente con una sua delegazione. Sarebbe utile in questa occasione che il Parlamento discutesse delle reali condizioni di vita e di lavoro nel Paese.

vedere di fronte alla fabbrica la scritta: «La Torino operaia vi piange», non per isolarsi dalla città ma per rivendicare quella condizione di lavoro produttivo su cui si basa una moderna società sviluppata come la nostra. Eppure, dentro quella fabbrica non c'erano squadre antincendio; c'era un superamento dell'orario di lavoro

per riconquistare uno spazio della loro vita; c'era uno straordinario consolidato (due di quei lavoratori sono morti alla dodicesima ora del loro lavoro e e succedeva spesso che arrivassero alla sedicesima ora di lavoro perché l'organico non era sufficiente). Non si possono sottacere le reticenze che ha incontrato la Commissione da parte, per esempio, dell'Azienda sanitaria, né le superficialità degli enti preposti al controllo: difatti l'INPS, a seguito di una ispezione, rileva che i contributi sono regolarmente versati - ci mancherebbe altro - e non invece che quei lavoratori sono costretti allo straordinario

in un'azienda ad alto rischio, che aveva subito 35 prescrizioni. Vorrei ricordare il procuratore della Repubblica che denuncia scarsi controlli, scarsa qualità dei controlli e - ancora peggio - una commistione tra chi controlla e chi ha consulenza dentro le aziende.

conto. Eparlare di questo non è parlare di altra cosa dal Protocollo. Avete visto le facce di quei giovani lavoratori, tutti trentenni, tutti entrati dopo il 1996, tutti a sistema contributivo e con montante contributivo;

Vorrei sollevare un altro punto. Questo accordo considera concluso il compromesso tra movimento operaio, capitale e Stato, quel che abbiamo chiamato il *welfare* *State* e che ha rappresentato il punto più alto in termini di intelligenza del rapporto tra democrazia e capitalismo e tra Stato e mercato, con una idea di funzione riequilibratrice attraverso una redistribuzione delle risorse.

sposta aree di decisione di interesse generale dalla politica all'impresa. È cioè quella la radice dell'antipolitica. Possiamo dire, da notizie certe, dall'intervento pesante di Confindustria, anche in rapporto alle modifiche apportate alla Camera, che c'è uno spostamento dall'area della politica di quella concezione politica riformatrice che aveva accentuato la sua pressione sul capitalismo. Oggi il compromesso su cui si basava quel keynesismo favorevole all'intervento pubblico a sostegno della domanda e sulla redistribuzione delle risorse subisce quell'offensiva, come la chiama Giorgio Ruffolo, cavalca la riscossa del pensiero neoliberista, respinge l'intervento dello Stato nel mercato e ha la fiducia indiscussa nella capacità di autoregolazione dello Keynes disse un giorno che non era lontana l'epoca in cui far denaro sarebbe stata considerata una delle più turpi patologie dell'anima.

ha subìto quella offensiva capitalistica abbia distrutto il tessuto industriale del nostro paese. Penso all'industria aerospaziale e ai cantieri navali, per non parlare dell'Alitalia

Sono sotto gli occhi di tutti le polemiche ai più alti livelli istituzionali. Questo appunto perché

È una vicenda di politica della concertazione. È evidente che il Governo ha assunto impegni senza avere una maggioranza politica.

programmatiche significative e si ristabilisca una connessione sentimentale con il Paese e le sue condizioni reali, oppure dovremo trarne le conseguenze.

Vorrei parlare però della parte più rilevante di questo accordo, che è la normativa in materia di accesso al pensionamento anticipato. È evidente che, da questo

Ma non c'è dubbio che, nel complesso e a regime, questo accordo alza l'età pensionabile e diminuisce i rendimenti delle pensioni. Non è mai accaduto,

agisce sui giovani - come ho poc'anzi ricordato - assunti dopo il 1996, abolendone in sostanza la pensione di anzianità, diminuendo il montante contributivo con gli sgravi

le donne nel loro diritto alla pensione di anzianità. Sembrava che in questo Parlamento si fosse formata una maggioranza trasversale, che tenesse in considerazione la famiglia. Come se queste famiglie non fossero rette dal lavoro di cura, di produzione e riproduzione sociale delle donne. In questo Paese, le donne andavano cinque anni prima in pensione, rispetto agli uomini, appunto perché il compromesso sociale del movimento operaio individuava in quel lavoro di cura, di produzione e riproduzione sociale la necessità

la fine di un compromesso socialdemocratico. Il Governo, senza avere una maggioranza politica, ha definito un'intesa con il sindacato: credo che sia stato un ampio esercizio di democrazia, ma di una democrazia,

con questo accordo finisce una fase politica. Ci auguriamo che, a partire da una riflessione sul lavoro e sulla sua condizione in questa società, si possa riaprire una fase politica che riconnetta azione di Governo e

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, gli interventi dei senatori Brutti Paolo e Zuccherini

entro cui questa vicenda si inserisce: una situazione di totale solitudine e di deprezzamento del lavoro operaio che dura da tempo e che forse avrebbe avuto bisogno, da una coalizione e da un Governo di centro-sinistra, di segnali di inversione di tendenza molto più netti di quelli che sono arrivati nel corso di questo anno e mezzo Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad un accordo, e quindi ad una normativa che lo traduce in legge, che per tanti aspetti è discutibile ed è stato molto discusso nel corso di questi mesi. Già si è detto dei meccanismi di compensazione interna, del passaggio dallo «scalone» di Maroni agli «scaliniۚ» di questa legge che di fatto, a fine percorso, aumenta l'età pensionabile per le pensioni di anzianità. Nasce la preoccupazione che le misure, troppo limitate nell'incidenza e nel ventaglio, relative al mercato del lavoro stiano ad indicare un intervento su queste materie che praticamente si lascia alle spalle l'intento presente nel programma dell'Unione di superamento della legge n. Restano aperti, infatti, problemi molto importanti: mi riferisco ad una diversa normativa relativa alla cessione del ramo d'azienda, che sta diventando il principale strumento di smantellamento dei diritti acquisiti di settori importanti di lavoratori; mi riferisco ad una questione che non viene mai sufficientemente discussa, cioè del rapporto tra pubblico e privato nella gestione del collocamento così come definita nella legge n. 30, che che crea sovrapposizioni e forme di privatizzazione estreme e che, tra l'altro, non aiuta a definire una distinzione di ruoli che sarebbe necessaria tra il pubblico e il privato nella ricostruzione di un mercato del lavoro contrassegnato dall'equità e dalla trasparenza. Naturalmente adesso sarebbe ingiusto e sbagliato, soprattutto rispetto al nostro Governo e alla maggioranza che lo sostiene, non sottolineare gli aspetti positivi che sono contenuti in questo testo. Mi riferisco alle misure relative alla totalizzazione dei contributi; all'aumento, anche se relativo, delle pensioni minime; all'intervento sull'indennità di disoccupazione.

però, non mi sembra questo il problema rilevante. È che nella discussione parlamentare - come è stato sottolineato con forza dall'opposizione

sostanza, è stato arrecato un *vulnus* alle prerogative parlamentari con il disconoscimento da parte del Governo del lavoro fatto dalla maggioranza nella Commissione bilancio della Camera,

Il presidente Treu ha detto in più occasioni - da ultimo questa mattina - che, quando ci si trova di fronte ad accordi concertativi, vi è sempre una certa forzatura della volontà parlamentare.

e funzioni parlamentari, nella relazione stretta tra attività parlamentare e relazioni sociali, esistono sempre questioni aperte che riguardano il merito e le procedure.

Governo: in questo accordo di concertazione mai come prima non vi è stato scambio tra le parti, né tra il Governo e le parti sociali. Credo che questo sia l'indice del fatto che ci troviamo di fronte ad una concertazione *sui generis*. In sostanza, ci troviamo di fronte al fatto che il Governo ha sottoposto - e aggiungo: giustamente - alle parti sociali una materia che era sua esclusiva esclusiva prerogativa, o meglio esclusiva prerogativa del Governo e del Parlamento. L'ha sottoposta ad una consultazione delle parti sociali per trovare il loro consenso.

la consultazione dei lavoratori, visti gli esiti della discussione parlamentare, può divenire un altro degli elementi di involuzione plebiscitaria della democrazia del nostro Paese.

del Governo nei riguardi del Parlamento di fronte ad accordi concertativi, ha sempre avuto una soluzione. La maggioranza parlamentare che sostiene il Governo si è fatta garante delle procedure parlamentari che stanno alla base degli accordi concertativi. Io mi chiedo - e me lo chiedo ancora dopo mesi - per quale motivo

al rapporto con le parti sociali per definire la piattaforma con cui arrivare alla discussione parlamentare. Questo mi pare uno degli elementi che va anche al di là dei problemi della vicenda politica a cui si riferiva il collega Zuccherini, e cioè della necessità di una verifica politica. Mi pare un aspetto delicatissimo quello di questi, diciamo, snodi critici della nostra vita democratica che debbono trovare, da parte del centro-sinistra e da parte di tutte le forze politiche, un'adeguata soluzione in avanti. A proposito della verifica di Governo che è stata ampiamente annunciata dalle forze di sinistra, però, io credo che un problema si ponga anche per noi, per le forze della Sinistra Arcobaleno che già in alcune occasioni ha avuto modo di intervenire a questo titolo e con questo nome nella discussione politica e parlamentare in quest'Aula. Mi riferisco al fatto che dietro questa vicenda vi è una questione mai affrontata esplicitamente nel suo rapporto con il resto della maggioranza da parte dell'intera sinistra, e quindi da parte di noi stessi. Dietro questo problema esistono delle scelte di politica macroeconomica che riguardano i problemi relativi alla gestione del debito che, nel corso del dibattito politico di questi anni e nelle scelte di Governo, nel modo che sappiamo da parte del Governo e soprattutto da parte del Ministro dell'economia, in ossequio alle indicazioni che venivano dall'Unione Europea, con una sostanziale proposta di sterilizzazione del debito da parte di alcuni economisti della sinistra; ma vorrei dire che, da parte di noi, che abbiamo la responsabilità politica e parlamentare della gestione della questione, io credo che sia stata sostanzialmente la sottovalutazione di un intervento specifico e di una posizione specifica su questo tema. Ciò ha consentito ai nostri avversari politici, e qualche volta anche ai nostri alleati, di presentarci semplicemente come un irresponsabile partito della spesa. No, noi non siamo questo: siamo una forza che vuole avere un profilo ed uno spessore di forza di Governo, e quindi probabilmente, in vista della verifica che andremo a fare a gennaio, su questo dobbiamo elaborare una nostra specifica posizione;

Insomma, io credo che il prosieguo di questa discussione sia anche una sfida per noi e io sono fiducioso del fatto che la sapremo affrontare nella maniera migliore, sia nel dibattito politico che nel prosieguo della vita del nostro Parlamento.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento in discussione, frutto di un faticosissimo e farraginoso confronto fra le parti sociali e il Governo, è molto, molto distante dall'esigenza di dare risposte vere e credibili al malessere sociale ed alla condizione oggettiva di milioni di lavoratori e lavoratrici, giovani e pensionati, che vivono drammaticamente la loro condizione salariale e sociale e non ce la fanno più ad arrivare a fine mese, come le statistiche più volte pubblicate sui giornali ci evidenziano. La condizione salariale dei lavoratori italiani è l'ultima in classifica a livello europeo (naturalmente nell'Europa a 15), sia per quanto riguarda quello che gli industriali chiamano il costo del lavoro, cioè il salario lordo, sia per quanto riguarda il salario netto. Inoltre, mentre i salari negli altri Paesi europei, negli ultimi cinque anni sono aumentati notevolmente oltre i livelli di inflazione, i nostri hanno perso potere d'acquisto. I contratti nazionali di lavoro non si rinnovano, la media di ritardo è di undici mesi (a questo proposito è emblematica la situazione della FIOM) ed a stento garantiscono il potere d'acquisto dei salari stessi. Vivono in una condizione di precarietà e sottosalario milioni di giovani, a cui è stata tolta la possibilità di programmare il futuro.

perché io sono stato meglio di mio padre, mio padre è stato meglio del suo e così andando indietro nel tempo. Oggi i nostri figli hanno davanti a loro la prospettiva di stare peggio dei loro genitori, non solo dal punto di vista salariale ma, più in generale, rispetto ai diritti e alle loro libertà. alla precarietà del rapporto di lavoro, sui giovani pesa ancora più forte la condizione salariale, che mediamente oscilla tra i 500, 600 euro ai 1.000 - per i più fortunati - al mese; mentre nel resto d'Europa mediamente i lavoratori precari percepiscono il 30 per cento in più di salario rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato,

E questa condizione di precarietà - badate - è destinata ad aumentare proprio perché, se non si affronta contemporaneamente la piaga del sottosalario, è fuor di dubbio che i datori di lavoro saranno sempre di più incentivati ad assumere lavoratori precari perché costano di meno. È una condizione inaccettabile che questa maggioranza si era impegnata nel suo programma a superare, così come era previsto il superamento del famigerato scalone Maroni, che a partire dal 1° gennaio 2008 elevava a 60 gli anni necessari per l'accesso alla pensione di anzianità per tutti. disegno di legge in questione è frutto di un accordo di concertazione fra le parti sociali ed io non voglio sottacere o dire che al suo interno non vi siano anche elementi positivi, soprattutto rispetto ai giovani (penso alle misure di incentivazione per il lavoro, al riscatto delle lauree, al ricongiungimento dei periodi assicurativi e così

che permettono l'accesso al pensionamento anticipato di tre anni, ai lavoratori appunto soggetti a mansioni e a turni particolarmente usuranti. Un altro punto critico è quello relativo alla precarietà, dove si afferma la possibilità per le imprese di reiterare dopo trentasei mesi il rapporto di lavoro in deroga al tetto, senza definire i limiti massimi di tale rinnovo. A questo proposito voglio sottolineare che la direttiva europea prevede che il tetto massimo di ricorso al lavoro a tempo determinato sia di ventiquattro mesi. In particolare, su questi due temi alla Camera si erano individuate soluzioni migliorative che, non stravolgendo né l'accordo né il disegno di legge, miglioravano lo spirito dell'accordo stesso. L'accordo raggiunto in Commissione lavoro alla Camera non è stato frutto né di ricatti né di imposizioni, ma dettato unicamente da regole di buon senso condivise anche dal Governo, a partire dal Ministro dell'economia e delle finanze, che è stato lungamente presente nel confronto parlamentare. Nell'Aula poi è accaduto un fatto gravissimo, come già sottolineato da altri miei colleghi: su pressione della Confindustria e anche di alcune parti del sindacato, ma soprattutto sotto il ricatto di alcuni esponenti della nostra maggioranza qui al Senato, che in nome del rigore e del contenimento della spesa hanno minacciato di non votare il provvedimento, il Governo ha posto la fiducia su un maxiemendamento che ha cancellato parti importanti e qualificanti del provvedimento mortificando così l'autonomia del Parlamento e dando uno schiaffo sociale ai lavoratori precari e agli altri lavoratori che si sono visti scippare la possibilità del riconoscimento di un loro sacrosanto diritto dopo anni di lavoro particolarmente usurante. Tra l'altro, si tratta nella maggior parte di casi di lavoratori cosiddetti precoci, cioè di lavoratori che hanno iniziato la loro vita lavorativa tra i quindici ed i Inaccettabile poi è stata questa operazione del Governo, il ricatto rispetto all'autonomia parlamentare. Già altri si sono dilungati al riguardo; io voglio solo ricordare che non siamo uno Stato corporativo: l'autonomia del Parlamento deve essere comunque garantita e non possono valere i ricatti di nessuno.

le regalie, le rendite di posizione e di potere dei ceti e delle classi più abbienti, che in questi anni hanno visto aumentare la loro parte di reddito disponibile a scapito dei lavoratori, che invece si sono visti tagliare Stato sociale, salari, pensioni, a fronte di un aumento vertiginoso dei prezzi e delle tariffe. Ritengo poi che da parte di molti sia un po' farisaico,

accade quel che è accaduto a Torino; quando la politica e le istituzioni si sono presentate

della precarietà, la questione della sicurezza sul lavoro non potrà essere affrontata. Se non c'è sicurezza del lavoro, è impensabile garantire la sicurezza sul lavoro.

dall'altra, siamo il Paese che ha il primato del più alto numero di infortuni e del più alto numero di infortuni mortali in Europa: un milione di infortuni ed oltre 1.000 morti anche quest'anno, con un costo sociale a spese delle casse dello Stato, oltre al dolore che si crea nelle famiglie, alla perdita di vite umane,

Il terzo elemento è la produttività del sistema Italia in caduta libera, che spesso, soprattutto da parte della Confindustria, viene invocata per andare a un'ulteriore stretta sui salari e sull'aumento delle prestazioni. Non si parla mai di produttività del lavoro: la produttività del lavoro in Italia, oltre a quanto ho già detto sul costo del lavoro, è tra le più alte d'Europa. la produttività del sistema ad essere tra le più basse ed è in caduta libera. Questa perdita di produttività, a mio parere, è la conseguenza di un errore pervicacemente continuato, in particolare dalle nostre controparti, e assecondato sia dal sindacato che dalla politica, che per affrontare e risolvere i problemi della produttività sia sufficiente intervenire sul costo del lavoro. Bassi salari, pochi diritti, alta precarietà non favoriscono l'aumento di competitività del sistema Italia, mantengono per un periodo transitorio alto il profitto, ma portano al declino

sul costo del lavoro e ulteriori aumenti di flessibilità. Trovo poi singolare la posizione della Confindustria, che si associa alla denuncia che ultimamente ha fatto notizia su tutti i giornali, sul fatto che in Italia esiste una questione salariale, che pensionati e lavoratori non ce la fanno più, che i salari sono troppo bassi, che ciò ha effetti negativi anche sulla domanda di beni primari e poi, contemporaneamente da una parte oppone resistenza sui rinnovi contrattuali e dall'altra pensa che la soluzione per l'aumento dei salari dei lavoratori debba essere trovata prendendo i soldi dalla tasche dello Stato. dunque, se in Italia i salari sono bassi la colpa non è di una politica economica redistributiva salariale

Stato. C'è oggettivamente un'ingiustizia, una pressione fiscale troppo elevata che va affrontata: in questo senso nel disegno di legge finanziaria abbiamo già deciso che le prossime disponibilità finanziarie entrate dovranno essere destinate ad una riduzione della pressione fiscale sui lavoratori dipendenti. Però,

di merito sul provvedimento rimane complessivamente negativo. Si poteva e si doveva migliorare; se il Governo porrà la fiducia, noi la voteremo per coerenza e per il fatto che, se non la votiamo, c'è il ricatto del ripristino del cosiddetto scalone Maroni. la fiducia non perché modifichiamo il giudizio sul provvedimento, ma perché la vostra azione è più complessiva rispetto all'operato del Governo, che su altri provvedimenti abbiamo apprezzato, e soprattutto è necessaria alla sua sopravvivenza.

Dopo la finanziaria si deve dar luogo ad una verifica e ad un confronto vero e si devono individuare alcuni punti fondamentali sulle questioni sociali: la questione salariale,

all'attenzione due elementi che cercherò di non ignorare, pur nella ristrettezza e nello schematismo di un intervento che deve avere una durata assolutamente limita.

Abbiamo sentito definire il programma dell'Unione roba da archeologia industriale; abbiamo sentito

Ad esempio, quando si giudica l'operato delle rappresentanze sociali e si esprimono le valutazioni che abbiamo ascoltato sulla concertazione, se penso ad altri periodi della storia di questo Paese, spesso quelle stesse osservazioni erano formulate dalla destra, piuttosto che dalla sinistra: dire, cioè, che il Parlamento viene sottoposto «prendere o lasciare», un accordo concertato tra Governo e parti sociali, era una critica che eravamo abituati a sentire da altre parti politiche piuttosto che dalla sinistra, come invece abbiamo ascoltato in questa circostanza. Mi interrogo anche sulla novità e sul giudizio di rappresentatività che ho ascoltato, e che continuo a sentire, durante questa discussione sul livello di rappresentatività del mondo del lavoro, delle organizzazioni sindacali, persino quando coinvolgono in un giudizio 5 milioni di lavoratori in carne ed ossa, uomini e donne che si recano a votare ed esprimono un giudizio con il loro voto sul contenuto di questo accordo. Penso che ci sia sufficiente materia non solo per analizzare politicamente la conclusione di questa fase. Spero che non sia la conclusione di un'alleanza politica e che quindi ci siano le condizioni perché l'attività della maggioranza che ha vinto le elezioni possa proseguire nel corso di questa legislatura. Probabilmente dovremo anche confrontarci e interrogarci sul livello di rappresentatività che le forze politiche, il Governo e le parti sociali sviluppano nel corso della dinamica della difesa degli interessi, che, mi pare di capire, in questo momento è fortemente in discussione per le modalità con le quali si è sviluppata finora. Ho sentito parlare il collega Di Siena di una sorta di rafforzamento del metodo plebiscitario, sviluppato dai sindacati che propongono l'approvazione di un accordo che hanno sottoscritto. Non ho trovato niente di nuovo nelle modalità che normalmente i sindacati seguono anche quando firmano un contratto di lavoro: lo firmano e poi si riservano, come sempre, di sanzionarlo in via definitiva, dopo un'ampia consultazione della parte che rappresentano. Vorrei che

forse più figlia della tensione, del confronto e anche dello scontro politico che si è sviluppato nel merito, piuttosto che valutazioni più generali su come il sistema politico e il sistema rappresentativo nel nostro Paese si stiano evolvendo nel corso di questi anni. Quanto al secondo punto, che riguarda il merito, non vorrei semplificare concetti che sono complessi e che probabilmente chi segue le vicende lunghe della previdenza, e ha seguito in questi anni diversi provvedimenti di riforma, a partire da quello principale che ha innovato, ossia il provvedimento che passa sotto il nome di riforma Dini, sa quanto abbiano interessato il confronto su questa materia. esemplificare per sostenere che mi pare che non ci sia discussione sul fatto che vivere più a lungo, come abbiamo registrato essere il dato con il quale ci dobbiamo misurare, costa di più, costa di più, soprattutto se noi, il centro‑sinistra, vogliamo che questo vivere di più si realizzi sempre in una società che mantiene il suo carattere solidale. se vivere di più costa di più, ciò significa anche avere la consapevolezza che occorre aumentare la platea di chi contribuisce a garantire con il con il suo contributo proporzionato una società solidale. Il tema con il quale ci siamo misurati in questi anni, ossia l'aumento dell'età per concludere la carriera di lavoro, in fondo è questo.

Ho sentito parlare spesso di modelli scandinavi, dimenticandoci che lì esiste una platea di popolazione che è cinque o, in qualche caso, anche dieci volte inferiore a quella che caratterizza Paesi della dimensione

del tasso di attività non di gente che è occupata o disoccupata, ma che è disponibile a lavorare. È un concetto profondamente diverso, che ho colto anche nell'intervento del senatore Viespoli, che forse non è stato colto del tutto, quando ha detto che il problema lo risolviamo pensando al Mezzogiorno. Certo il Mezzogiorno contribuisce, ma anche il tasso di disponibilità a lavorare della parte più sviluppata del nostro Paese

rispetto a quell'obiettivo di aumentare la platea di chi contribuisce a garantire equità in una società solidale come quella che noi vogliamo realizzare. In questo contesto,

a migliorare, a cambiare ciò che è necessario e indispensabile modificare, affinché questa nostra società mantenga quei caratteri di solidarietà, di coesione che abbiamo cercato di salvaguardare nel corso degli anni che ci lasciamo alle spalle,

da questo punto di vista il fatto che ci siamo proposti l'obiettivo di evitare che in una notte l'età pensionabile facesse un balzo va inquadrato in un contesto nel quale noi riaffermiamo e confermiamo l'obiettivo di graduale e stabile innalzamento dell'età della pensione (perché a questo non possiamo, evidentemente, rinunciare), ma cerchiamo di farlo in maniera più equa e contemporaneamente accompagniamo a questo provvedimento una serie di altri, fra i quali quello relativo al tema dei cosiddetti lavori usuranti. Mi permetto di dire che non sempre l'ho sentito trattare

avendo un'aspettativa di vita mediamente inferiore, si giustifica il fatto che la sua conclusione del periodo lavorativo, sempre per un principio di equità, sia inferiore a quella della media generale, proprio perché chi è impegnato in un lavoro usurante è statisticamente dimostrato che è sottoposto ad una vita di lavoro più nociva e quindi ad un'aspettativa di vita inferiore. Per questa ragione, l'individuazione di questa categoria di lavoratori deve essere fatta con molto rigore e con particolare attenzione, perché le motivazioni per le quali noi riconosciamo a questa categoria di lavoratori un accorciamento

nell'allargare questa fascia (come spesso accade nella nostra discussione) stiamo producendo, per così dire, un danno, stiamo commettendo un'ingiustizia nei confronti di quella fascia di lavoratori che effettivamente corrispondono a questa attività.

non stabiliamo che il Governo, nel momento in cui tratta con le parti sociali i contenuti della concertazione, verifica preliminarmente, sotto il profilo dell'indirizzo, quali sono i limiti e le compatibilità del mandato che gli viene assegnato, rischiamo effettivamente di vanificare la concertazione. Io ho questa impressione. Da questo punto di vista è chiaro,

mal utilizzata, perché il Governo, se ha una sua maggioranza politica, così come quando sigla trattati di carattere internazionale che in questa sede ratifichiamo senza discutere, deve avere l'autorevolezza di poter stipulare anche accordi di questa natura. In conclusione,

che dobbiamo continuare a seguire, applicando sempre più coerentemente il principio di equità, che è uno dei punti fondamentali del nostro programma di Governo (che spero nessuno lo consideri archeologia industriale), ulteriormente migliorando ed adeguando ogni misura che riguarda il sistema del *welfare* e in particolare il lavoro e la condizione delle generazioni più giovani: dalla previdenza, al diritto alla formazione permanente, alla flessibilità - che non è una parola negativa - mai separata dai diritti e dalla dignità del lavoro, valore in sé, a prescindere dai vincoli di mercato. Credo che, se resteremo fedeli a questi principi, continueremo a migliorare la condizione generale

il professor Giulio Tremonti, dieci anni fa, scrisse un libro anticipatore e nello stesso tempo profetico,

alla globalizzazione e alla grande trasformazione che era in corso. Quali sono state le conseguenze di quell'opzione?

G8. In quegli anni - ma anche ora - nei banchi della sinistra si parlava della solidarietà, dell'immigrazione: non a caso,

cento. Quando studiavamo economia politica all'università ci hanno insegnato infatti che, quando aumenta l'offerta, i prezzi scendono; quindi, il costo del lavoro scende.

diminuisce l'IRES dal 33 al 27,5 per cento. Cosa scrive un intellettuale di sinistra onesto sul «Corriere della Sera» del 24 ottobre scorso? Che la politica di centro-sinistra favorisce la grande impresa settentrionale e le banche.

verso il salario operaio, verso i redditi del ceto medio, non hanno mai attuato una politica diversa da quella che stanno realizzando. Voi avete

Con il pacchetto Treu non stabilizzavate nulla: avete utilizzato la riforma Biagi per stabilizzare i lavoratori. La vostra riforma, quella del centro-sinistra, creava centinaia di migliaia di precari a vita con i Co.co.co., i collaboratori coordinati e continuativi.

viene riattivato)*... 4 milioni di italiani vivono di lavoro nero. Questa è la sinistra di Governo, questa è la sinistra bancaria che in realtà fa gli interessi del turbocapitalismo.

cercherò di fare una rapida ricostruzione degli eventi di questi giorni con una breve premessa, cioè che tutti gli argomenti che sono stati discussi nelle ultime ore, che hanno formato l'oggetto della proposta che il Governo ha avanzato alle associazioni e che hanno fatto sì che quella parte di associazioni che aveva proclamato il fermo lo abbia ritirato erano già ampiamente in discussione fin dal mese di febbraio di quest'anno, quando fu sottoscritto un protocollo d'intesa il Ministero dei trasporti e le associazioni di categoria, fatta eccezione per la Confartigianato e per il FAI. Quel protocollo prevedeva una serie di impegni che il Governo avrebbe dovuto affrontare, sia sul piano normativo che sul terreno finanziario, per andare incontro alle esigenze esposte dalle associazioni stesse. L'attuazione di questo protocollo è stata seguita con riunioni mensili tra la Direzione generale dell'autotrasporto del Ministero e le associazioni stesse per verificarne, strada facendo, lo stato di attuazione.

dei punti che erano stati indicati erano già risolti. Ne rimanevano ovviamente altri, per alcuni dei quali si stavano predisponendo apposite misure nella finanziaria 2008, attualmente in discussione.

hanno dichiarato l'inconsistenza dell'azione svolta dal Governo da febbraio fino a novembre per affrontare i problemi che ho accennato e, conseguentemente, dichiaravano la loro intenzione di proclamare un fermo che sarebbe stato poi successivamente formalizzato il 14 novembre da due di queste associazioni, la FITA-CNA e la Confartigianato.

comportati dalla crescita esplosiva negli ultimi mesi del prezzo del gasolio, crescita che ovviamente ha avuto una ricaduta diretta sul costo di esercizio dell'autotrasporto e per la quale è stato chiesto l'intervento governativo.

produttive, competenti in materia, che si poneva questo problema e chiedevo di studiare una soluzione nell'ambito delle compatibilità della normativa europea. In sostanza, non si dovevano configurare come aiuti di Stato. Rispetto alla proclamazione del fermo, in data 20 novembre, ho provveduto a convocare tutte le associazioni per il giorno 23, attuando attuando quella che viene normalmente definita la procedura di raffreddamento per tentare di trovare una composizione. Ma le associazioni che avevano programmato lo sciopero, insieme alla FAI e ad altre, hanno dichiarato la loro indisponibilità a partecipare alla

All'inizio di dicembre, unitamente al sottosegretario Letta che ha seguito sempre molto da vicino la vicenda, ho convocato tutte le associazioni per discutere in quella sede i problemi sollevati dalle due associazioni che avevano proclamato il fermo. Poiché hanno insistito per chiedere un tavolo separato, la riunione è continuata nonostante esse abbiano abbandonato la seduta

che portano merci ritenute di stretta necessità, come l'approvvigionamento di materiali agli ospedali e del carburante in genere.

che erano in corso forme di manifestazione all'interno di quello che veniva definito un fermo che erano veri e propri blocchi della circolazione. Generalmente le

Questa situazione non poteva comunque essere accettata, perché non solo non rientrava nell'ambito del codice di autoregolamentazione, ma ricadeva addirittura nella fattispecie della violenza privata

Questo è il motivo per cui alla fine ci siamo determinati, in accordo con la Presidenza del Consiglio, per emanare un'ordinanza che impropriamente è stata chiamata di precettazione, la precettazione è un meccanismo che si applica nel caso dei servizi pubblici, nei confronti degli operatori del servizio pubblico. In questo caso, l'ordinanza stabiliva l'arresto del fermo stesso, della manifestazione stessa, a partire dalla mezzanotte di martedì. Ovviamente abbiamo dovuto, a seguito dell'ordinanza, chiedere al Ministero dell'interno e alle prefetture di disporre la presenza sulle strade delle Forze dell'ordine per assicurare il rispetto dell'ordinanza stessa. Nella giornata di mercoledì l'effetto dell'ordinanza e della presenza delle Forze dell'ordine aveva leggermente ma progressivamente allentato la presa di queste situazioni, soprattutto nei punti più caldi, era evidente che avremmo avuto diverse altre giornate di grande difficoltà. Questo è il motivo per cui, parallelamente, abbiamo chiesto di nuovo alle associazioni tutte assieme, comprese quelle che avevano proclamato il fermo, di tornare a discutere su quale poteva essere una base di intesa perché venisse revocato in via ufficiale, e non solo contrastato con la nostra ordinanza,

insieme al sottosegretario Letta, abbiamo consegnato a tutte le associazioni una proposta del Governo che era sostanzialmente una messa a punto del vecchio protocollo d'intesa integrato con alcune delle richieste che erano state avanzate negli ultimi giorni, in modo particolare quelle relative alle modalità con cui sterilizzare in qualche modo i costi insorgenti dall'aumento del prezzo del gasolio.

anche queste ulteriori parti rispetto al protocollo d'intesa di febbraio a condizione che venisse rimosso il fermo.

da quell'ora, la situazione si è rapidamente stabilizzata. Direi che, ad oggi, a stasera, a quest'ora in cui siamo, si è completamente risolta

ma contemporaneamente di apertura al dialogo che abbiamo praticato, ha fatto sì che si recedesse da questa forma di protesta che, ripeto, era rapidamente degenerata.

che sarà sancita con un tavolo tecnico che avvieremo subito dopo la pausa di fine anno e con il quale contiamo di fare un'operazione analoga a quella che abbiamo appena condotto in porto per il trasporto pubblico locale, intendo dire l'emanazione di un vero e proprio progetto di riforma complessiva del settore dall'autotrasporto, che nel caso del trasporto pubblico locale ha trovato spazio nel disegno di legge collegato alla finanziaria. Credo realisticamente che nei primi 6-8 mesi del prossimo anno lo potremo mettere a punto, evitando così, com'è stato fatto nell'altro caso, che anno per anno si dovessero mettere a disposizione risorse per coprire esigenze che si rincorrevano sempre, affrontando una volta per tutte il il tema di fondo di questo settore che poi è quello della ristrutturazione aziendale. Questo è un settore in cui la stragrande

non vi è la capacità di contrastare un fenomeno, quale quello del lavoro nero, sottopagato, non coperto da previdenze sociali che singole persone provenienti molto spesso da da Paesi dell'Est o della riva Sud del Mediterraneo offrono, mettendosi alla guida di un camion posseduto da tutt'altro titolare.

Signor Presidente, ringrazio il Ministro per l'informativa puntuale e molto utile rispetto ad un fatto che ha allarmato e creato disagi disagi alla cittadinanza. A me pare che le questioni in ballo siano due: una attiene allo Stato di diritto in questo Paese; l'altra all'organizzazione del sistema dei trasporti nel nostro Paese e alle politiche di intervento pubbliche in questo settore. Riguardo allo Stato di diritto, esiste probabilmente un'immanente tendenza nel nostro Paese, che attiene probabilmente alla debolezza del processo costitutivo dello Stato unitario, a rispettare poco, poco, meno di quanto sarebbe utile e necessario, lo Stato di diritto. Rispetto a questo l'atteggiamento del Governo e della politica può essere di due tipi: il primo è di accondiscendere. un atteggiamento che abbiamo visto spesso, che porta ai condoni, agli indulti, alle sanatorie, alla tolleranza verso l'illegalità diffusa. Ma io credo che questo atteggiamento sia una delle parti del male dell'Italia. È quello che fa dell'Italia un Paese ormai arretrato sul terreno non solo dello sviluppo economico, ma anche civile; nega l'essenza stessa dello Stato liberale che consiste sostanzialmente nel rispetto dello Stato di diritto. L'altro atteggiamento, è quello di provare a correggere questa tendenza che pure sappiamo esiste nel nostro Paese, riducendo la tolleranza verso gli atteggiamenti di illegalità, assumendo con determinazione il rispetto del criterio dello Stato di diritto come elemento costitutivo del Governo del Paese. Da questo punto di vista - mi consenta, Ministro - ci aspetteremmo maggiore determinazione da parte del Governo. del Governo. Qualche giorno fa addirittura un prefetto della Repubblica invitava il sindaco di Roma ad aprire la trattativa con i tassisti che stavano bloccando la città. Non ho avuto notizia del fatto che il Governo sia intervenuto per correggere l'atteggiamento di quel prefetto. Mi aspetterei, a seguito dei fatti gravi avvenuti, qualche informazione su quante sono state le segnalazioni all'autorità giudiziaria, giudiziaria, le multe comminate, le patenti ritirate. Mi aspetterei con franchezza un atteggiamento più determinato dal Governo che sostengo in direzione della ricostruzione degli elementi essenziali dello Stato di diritto in questo Paese.

è l'ovvia conseguenza di un sistema organizzato su piccole imprese, sostanzialmente di natura precapitalistica. Quindi, abbiamo anche alti costi di trasporto, il che comporta anche costi delle merci tendenzialmente più alti che in altri Paesi e difficoltà di competere per le nostre imprese.

sciopero). A quel punto lo Stato interviene in qualche modo e lo fa riconoscendo benefici. Abbiamo una lunga storia di benefìci, tra l'altro dichiarati illegittimi, come tutti sappiamo, dall'Unione Europea, che hanno generato a loro volta la necessità di provvedere, di sanatorie, poi dichiarate illegittime e così via. Ma sostanzialmente, alla fine, questa politica pubblica in cosa si manifesta? In meccanismi di incentivo. Ora, i meccanismi di incentivo cambiano le convenienze relative a favore del trasporto su gomma, quindi aggravano il problema dell'eccesso di trasporto su gomma. Sono meccanismi di incentivazione che cambiano le convenienze a favore di un'organizzazione precapitalistica, perché, in fondo, stiamo agevolando la piccolissima impresa, che in questo settore è particolarmente inefficiente e determina il 40 per cento di camion che viaggiano gratis, con gli effetti che ho detto. Quindi, sostanzialmente, una politica dell'intervento pubblico costretta permanentemente ad inseguire l'emergenza si traduce in una politica dell'intervento pubblico che contraddice le finalità che dovremmo perseguire: spostare il trasporto ad altri mezzi e favorire un riorganizzazione capitalistica. Mi auguro che anche su questo terreno, al di là del provvedere a fronte delle emergenze, si possa immaginare un ripensamento delle politiche pubbliche nel settore. PRESIDENTE. Signor Presidente, signor Ministro, le sue comunicazioni, o giustificazioni, su uno sciopero che ha coinvolto

o forse l'ora e il giorno sono stati fissati proprio per evitare un dibattito più completo, al fine quindi di evitare al Governo un'ulteriore figuraccia Aula? Signor Ministro, comprendo moltissimo il suo imbarazzo, perché certamente la sua onestà mentale avrà dovuto rilevare e avrà valutato l'inutilità totale della condotta del Governo di cui ella fa parte, considerando che, come titolava stamattina qualche giornale, il Governo è andato sotto i TIR

Vi siete accorti così tardi che mai come questa volta lo sciopero degli autotrasportatori era quasi un atto dovuto, perché il vostro Governo non aveva soltanto disatteso gli impegni legittimi assunti dal Governo Berlusconi, ma addirittura aveva negato agli autotrasportatori la possibilità di un semplice incontro. Lei parlava di incontri, ma di incontri inutili, perché poi quando avete voluto un incontro avete risolto tutto,

Chi ripagherà i disagi di milioni di italiani e i miliardi di danni subiti? Credo, signor Ministro, che qualunque risposta, o meglio, qualunque pezza che ella vorrà mettere alle sue comunicazioni odierne non potrà mai ripagare il disastro che ancora una volta ella e il suo Governo hanno provocato agli italiani. Certamente credo che abbiate valutato che le tardive concessioni, dovute, che avete fatto agli autotrasportatori valgono zero rispetto al danno che inutilmente gli italiani e tutta l'economia del nostro Paese hanno subito a causa della vostra assoluta irresponsabilità. Se non avevate la forza di resistere, dovevate iniziare subito le trattative e concedere subito quello che avete concesso. Si è parlato, signor Presidente, dei problemi dell'autotrasporto, che conosciamo, addirittura assegnando delle colpe alle imprese individuali. Io dico che sono proprio queste centinaia di migliaia di imprese individuali che consentono all'Italia di muoversi. Oggi non vi sono delle grosse organizzazioni nel settore dell'autotrasporto. Il Governo ha assolutamente evitato e annullato ogni politica dell'autotrasporto e queste sono state le conseguenze, signor Ministro. Oggi non vi è una politica dell'autotrasporto e mi fa piacere che lo abbia sottolineato anche il collega senatore D'Amico; avete assolutamente ignorato la situazione del Paese, e avete assolutamente ignorato, dando una prova di forza inutile, cento dell'economia del nostro Paese viaggia con gli autotrasportatori sulle autostrade. Allora, signor Ministro, credo che ella e il vostro Governo abbiate ancora contribuito a mettere, voi stessi, con il vostro ritardo, con la vostra irresponsabilità, il Paese in ginocchio. Grazie ancora a nome di tutti gli italiani, signor Ministro: avete veramente contribuito ancora una volta

nella giornata di ieri per porre fine ad una situazione estremamente preoccupante e grave, che aveva assunto anche alcuni connotati di rivolta. Sono dell' opinione che i problemi che si presentano in questo comparto siano estremamente gravi e che quindi bisogna seguirli passo passo, con attenzione e anche mettendo a disposizione delle risorse: a tale proposito suggerirò qualcosa nel mio intervento.

come tutti sanno, il punto centrale che la mobilitazione ha cercato di realizzare è stato quello della paralisi del trasporto della benzina e del gasolio.

e allora, per ottenere quel risultato, hanno utilizzato il sistema del blocco anche delle grandi imprese strutturate, delle autocisterne che trasportano il gasolio. Questi sono metodi di lotta che non rientrano nella tradizione di nessuna delle organizzazioni né sindacali, né autonome, né datoriali della storia del Paese. Se si imbocca questa strada si sa dove si comincia, ma non si sa dove si finisce. Detto questo, però, non c'è dubbio che le condizioni nelle quali si esercita questa durissima attività, questo durissimo mestiere, si sono aggravate anche repentinamente, perché non c'è dubbio che il costo del gasolio è cresciuto a dismisura, in modo estremamente rapido, il pedaggio delle autostrade che loro pagano, perché viaggiano sopra di esse, è altrettanto cresciuto in modo estremamente rapido e il processo di liberalizzazione del comparto è andato avanti a passi molto spediti, che non hanno tenuto conto della natura del comparto stesso.

a questo sciopero!), un settore, un comparto negozia con un Governo una serie di punti, sulla

Guardi, Ministro, che per guadagnare ciò che guadagna un autista del servizio pubblico, ad esempio dell'ATAC, che lavora meno di sei ore al giorno, gli autonomi devono lavorare almeno 15 ore al giorno. 15 ore al giorno. Poi ci si lamenta se succedono gli incidenti gravi, gravissimi o mortali. Queste sono conseguenze dell'incapacità di dare risposte. In un settore si usa una misura di un altro settore. Abbiamo capito che non amate il settore autonomo perché, secondo voi, tutto si deve strutturare in modo da essere concorrenziale su dinamiche di scala. Guardate che l'unica cosa che resiste in questo Paese sono gli autonomi. Appena un settore va in crisi, si chiude. L'autonomo non va mai in crisi; se va in crisi perché non guadagna, non farà altro che lavorare il doppio: non ha altra scelta se vuole stare sul mercato.

un Menenio Agrippa in grado di capire la complessità di questa società e di saper dare risposte armoniche ai tanti interessi che a volte confliggono in questo contesto.

l'avanzamento lungo una strada e su un terreno difficile. Credo di conoscere questo settore, anche se da 15 anni non me ne occupo più.

e con altri sindacati, vedeva l'amico Paolo Uggè dalla parte dei sindacati. La trattativa l'abbiamo fatta a Palazzo Chigi, come sempre di notte, perché le trattative degli autotrasporti hanno questa dinamica.

le organizzazioni che hanno tirato più di tanto la corda, abbiano deliberatamente promesso cose che si sapeva non si sarebbero potute ottenere dal Governo.

e credo che questo sia stato un errore, anzi un errore grave, perché ha fatto pagare alla categoria e al Paese un prezzo che non era giusto che pagassero. alla categoria e al Paese un prezzo che non era giusto che pagassero. Forse faceva parte della strategia della spallata, ma non si coinvolge una categoria di questo tipo in una strategia politica che non la riguarda.

dal modo di fare dei precedenti Esecutivi. Noi interveniamo meno sulla questione del petrolio, del gasolio, perché l'Unione Europea non ce lo consente più, però siamo alla ricerca di sostegni che favoriscano, in qualche modo, la sopravvivenza di questo settore così frammentato e rischiamo di tagliarne i fondi. Vorrei capire, per l'appunto, da dove vengano i 30 milioni destinati a coprire questo accordo, perché se provenissero da tagli al settore delle ferrovie (come sembra,

time* detta i tempi e i carichi di lavoro dell'autotrasporto e degli autotrasportatori. Ci accorgiamo che gli stabilimenti FIAT si fermano, ma non ne ricaviamo la conseguenza che a imporre quei ritmi e quelle condizioni sono le scelte organizzative dell'industria. Ci rendiamo conto che la direttiva Bolkestein e i processi di liberalizzazione a livello europeo ci scaricano grandissimi problemi dal punto di vista dei carichi di lavoro e della sicurezza. Ci dobbiamo rendere conto che o si

la descrizione che lei ci ha fatto, perché il 7 febbraio 2007 non un piccolo numero, ma la maggioranza delle associazioni dell'autotrasporto non hanno accettato il protocollo.

una volta dal suo capo di Gabinetto - per carità, sarà un'ottima persona - e in tale occasione e di concerto con le altre associazioni hanno richiesto risorse economiche pari a quelle definite nell'anno precedente, pari a 575 milioni di euro.

Nell'incontro tecnico di cui pure lei ha parlato del novembre 2007 il rappresentante del Ministro affermava testualmente che il Governo non poteva concedere ulteriori risorse rispetto a quelle previste nel citato decreto-legge decreto-legge e che gli impegni di protocollo dell'intesa del 7 febbraio 2007 venivano ulteriormente rinviati. Che deve fare una categoria, cari colleghi, quando

continuasse su questa strada, perché possono cambiare i Governi però l'impegno dello Stato verso una categoria va mantenuto. Quindi, non lesa maestà, ma semplicemente una categoria che in qualche modo è stata disattesa negli incontri: insomma c'è stato qualcosa di non corretto sotto il profilo dei rapporti istituzionali e sindacali. Questa è la realtà e, considerate le condizioni

provvedimento per la funzionalità del mercato e la normativa del settore, che interessa tutti quanti noi, e il problema dei controlli sulla strada, soprattutto con riferimento ai vettori esteri, l'introduzione del costo del gasolio in fattura, la previsione di un documento di tracciabilità per l'individuazione dei soggetti intervenuti nella filiera e la risoluzione di alcuni temi di carattere generale che già prima di me hanno ricordato.

lunghissimo sciopero degli autotrasportatori. Forse è per questo che il Governo di centro-sinistra, che ha tante responsabilità nella situazione generale del Paese, ha capito che c'era qualcosa di rivoluzionario in questo movimento.

ma alla saggezza della categoria che ancora una volta ha lanciato un messaggio al Governo e al Paese dicendo: abbiamo questi problemi, risolveteli.

minacciavano di non dare il loro sostegno in passaggi decisivi delle ultime settimane qui al Senato avesse posto fra le condizioni quella di dare qualche decina di milioni

che ne sono derivate per la popolazione, per il benessere dei cittadini e delle aziende, E nessun magistrato avrebbe pensato di indagare perché sono state fatte delle proposte politiche ad un senatore per assecondare le sue richieste, come invece capita in questi giorni al *leader* del mio partito che viene indagato per aver fatto politica, per aver fatto proposte politiche a dei senatori della maggioranza. Purtroppo, gli autotrasportatori non hanno trovato uno *sponsor* in un senatore che potesse minacciare di far cadere il Governo e dunque la cosa è stata completamente ignorata. Nel corso della distribuzione dei vari «tesoretti» accumulati nel corso dei mesi passati non si è pensato

che il prezzo dei carburanti è aumentato a dismisura negli ultimi mesi; sappiamo molto bene che le infrastrutture del nostro Paese sono in una condizione tale da mettere in grave difficoltà i nostri autotrasportatori; se poi pensiamo alle condizioni che trovano altrove, sia in termini di migliori infrastrutture sia in termini di tariffe assai più abbordabili (basta vedere quanto costa

a capire che le difficoltà dell'autotrasporto c'erano. Si sarebbero evitati i gravissimi danni di cui si è detto, che continueranno nei giorni a venire e che graveranno sulle spalle delle aziende, dei cittadini e del tessuto produttivo di questo Paese. Quanto ai problemi di ordine pubblico, certamente, come è stato sottolineato da senatori della maggioranza, non è ammissibile la violazione di leggi e bisogna tutelare lo Stato di diritto. Ma come mai ci si ricorda di questo solo a proposito di certe categorie, come i tassisti e gli autotrasportatori, quando per anni si è incoraggiato, tollerato, teorizzato il diritto di poche decine di persone, autonominatesi rappresentanti della loro categoria, di bloccare città intere con manifestazioni a volte autorizzate, a volte no? Evidentemente ci vuole una politica diversa, una politica che incoraggi le infrastrutture, che venga incontro ai lavoratori, alle aziende e ai comparti produttivi, come quello dell'autotrasporto, specialmente cercando di varare dei di varare dei forti sgravi fiscali. Il Governo Berlusconi ha lavorato in questa direzione, ma siamo ritornati alla vecchia tendenza, che ha privato il nostro Paese di infrastrutture per decenni, perché ci siamo concessi altri lussi, pagando le pensioni ai quarantenni, mantenendo molte persone a fare poco e

Lei ed il Governo, per affrontare il tema, avete cominciato a parlare di una nuova tariffa minima, di una serie di misure che dovrebbero regolare un po' la liberalizzazione, per salvaguardare la categoria

nel suo documento una serie di interventi importanti, intanto per abbattere i costi. Sono sicuro che una quota di risorse, che è stata recuperata

56 colleghi, non è più tollerabile che il tempo venga spesso male impiegato nelle aule elettive per discussioni del tutto estranee all'oggetto o per ostruzionismo. Il tempo è davvero denaro e nel nostro caso sono entrambi pubblici (scrivono i colleghi): si rendono quindi indispensabili modifiche sostanziali ai Regolamenti per contingentare al massimo i tempi di discussione e rendere rigido l'*iter* di esame dei provvedimenti in Aula e nelle Commissioni, al fine di evitare, nel rispetto di tutte le posizioni espresse, inutili divagazioni che allungano solo i tempi e rendono improduttivo il lavoro legislativo.

hanno scelto la settimana sbagliata. Se c'è stata una settimana nella quale l'ostruzionismo dei lavori parlamentari è stato compiuto dalla maggioranza e dal Governo, è stata questa. In questa settimana non abbiamo deliberato su nulla per la semplice ragione che

Ciò è inaccettabile, ma per l'opposizione, non per la maggioranza. La seconda considerazione, meno d'occasione e più, come dire, legata a quelli che sono i princìpi generali del nostro ordinamento e su cui le rivolgo una richiesta, è la da quando in qua 56 legislatori formulano alla Camera a cui appartengono una petizione? a disposizione uno strumento molto semplice: propongano una riforma del Regolamento, sviluppata per articoli, e la depositino formalmente. Ma evitino di utilizzare lei, signor Presidente, come terminale per un'iniziativa di carattere propagandistico

pratiche di carattere ostruzionistico. Ha sempre cercato, con gli strumenti del Regolamento, di far esplodere le contraddizioni esistenti nell'ambito della maggioranza, ma mai di andare al muro contro muro, come a lei è ben noto, signor Presidente, come lei ha più volte riconosciuto all'opposizione in questa Camera.

non per quanto viene additato come un problema dai 56 colleghi, tra i quali figurano molti valenti esperti dei lavori di quest'Aula,

da altri strumenti di cui non abbiamo davvero bisogno per comprimere ulteriormente la volontà del Parlamento. Quest'ultimo ha dimostrato in più di una occasione di saper deliberare, di saper tenere conto delle varie tesi anche in situazioni di forte contrapposizione che stanno caratterizzando l'attuale legislatura. Certo, bisogna dare modo come sta avvenendo in questi giorni - su un provvedimento non si può votare neppure una volta, è inevitabile che il Parlamento si esprima in modo conflittuale, con un muro contro muro, che si riduce ad una mera conta di voti che non è il lavoro che dovremmo svolgere.

oggi è stato ricevuto il Dalai Lama, prova di una grande sensibilità sua, Presidente, dei colleghi che hanno partecipato all'incontro di quelli e che l'hanno richiesto.

rappresaglie. La dignità delle istituzioni democratiche, la dignità di un Paese si mostra proprio facendo ciò che si ritiene giusto, anche se può - ma io ritengo che questo non avverrà - causare piccoli contraccolpi di carattere economico.